quando lei ieri non ci ha dato la parola dopo l'intervento del Governo è stato perché aveva stabilito di darcela oggi e di entrare nella discussione.

«Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale», considerato che:

sul quale però, non essendo pervenuta alcuna relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria, abbiamo dovuto confermare il parere contrario

una relazione tecnica positivamente verificata sull'emendamento 1.1500/5

Come da comunicazione che abbiamo appena ascoltato dal presidente Tonini, il quale ha confermato la presenza di una relazione tecnica e di un parere favorevole, confermo il mio parere favorevole. all'emendamento 1.127, del quale ho chiesto l'accantonamento per una verifica dopo la dichiarazione di inammissibilità di due subemendamenti,

si ritiene che l'emendamento 1.112, sul quale ho espresso parere favorevole con riformulazione, dia una risposta esauriente su questo tema.

81 della Costituzione per assenza di relazione tecnica, le chiedo l'autorizzazione a ripresentare una nuova riformulazione.

Grazie

la sanzione massima da 7.500 euro a 3.500 euro. Ora, mi rendo conto che nel mercanteggiamento con Forza Italia ci sia già l'espressione di un parere favorevole su un emendamento a prima firma della

e consigliare alla relatrice una maggiore prudenza. Sospendo la seduta fino alle ore 11 per dare modo alla Commissione bilancio di riunirsi.

A seguito della riunione della 5ª Commissione è stato espresso un parere, del quale do lettura: «La Commissione programmazione economica, bilancio, a revisione del parere precedentemente espresso sul subemendamento 1.1500/5, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

che prevede esattamente le cose che sono già nel nostro ordinamento. Mi rivolgo a lei, signor Presidente, per cercare di riportare un po' di razionalità.

Vorrei che tutta l'Assemblea - e lei ne è perfettamente a conoscenza - sappia che stiamo per votare una cosa che non modifica assolutamente nulla delle norme già esistenti. E tutto questo alle ore 11,20.

alla riformulazione dell'emendamento 1.0.1 (testo 4) sulle farmacie, che dovrebbe sostanzialmente confermare il punto di caduta del patto del Nazareno.

mi è dato sapere, risulterebbe ultroneo perché i minori sono già assoggettati alle norme sanitarie in vigore. Vorrei sottolineare una cosa: esiste forse una discriminazione, qualora dovesse essere posto in votazione questo subemendamento, tra i minori stranieri non accompagnati rispetto a quelli accompagnati,

di minori che arrivano nel nostro Paese ogni anno e che sono accompagnati. Per loro non valgono diritti o doveri in campo sanitario? Ve lo chiedo, colleghi.

Ieri mattina in Commissione bilancio, in maniera molto inaspettata e sorprendente, è arrivata la richiesta di coordinamento

se anche lei, Comandante, si ricorda: è stato quel giorno che abbiamo votato la sospensiva della sospensiva e poi la sospensiva. Dopo abbiamo parlato di tutto il coordinamento...

e quindi, ancorché ci separino delle divergenze di opinione, nessuno può abusare del tempo e della signorilità degli altri. altri. Dico questo perché ci troviamo di fronte ad un evento che non è trascendentale; è un patto tra il principale partito di maggioranza e il principale partito di opposizione.

poiché dura da ieri una manfrina su determinati subemendamenti, perché probabilmente è un subaccordo tra subindividui; non voglio crederlo, ma è tutto «sub». De Biasi).* Diciamo che è un accordo carsico. Perché non si ritirano i due Capigruppo insieme alla signora Ministro, che vediamo...

da Forza Italia perché io, Domenico Scilipoti Isgrò, rappresento Forza Italia e non ho fatto alcun inciucio né con il Partito

a livello europeo ed internazionale». Siccome su questo provvedimento aleggia l'ombra degli accordi presi nel 2014 da parte del Ministro (in una delle vostre classiche sessioni, in cui decidete sulla pelle nostra)

il Ministro ha deciso che l'Italia debba fornire i propri figli come cavie per sperimentare dodici vaccini, tutti insieme, sulla base di obblighi che non appartengono al popolo italiano, ma ad accordi presi oltretutto...

che venne poi allontanato della sua posizione in Aifa per un palese conflitto di interessi. Quindi, sinceramente, se dobbiamo stare agli obblighi del Ministro italiano, alzo le mani, ma se devo stare agli obblighi di altri trentanove Paesi, sinceramente ne faccio anche a meno.

Presidente, noi abbiamo presentato e votiamo questo emendamento. Qualcuno dice che non cambia le norme che già ci sono, però nelle norme già presenti c'è scritto che gli stranieri residenti sul nostro territorio, in particolare i minori, vengono iscritti al Servizio sanitario nazionale. Questo non è direttamente correlato al fatto che siano sottoposti ai medesimi obblighi. Noi di tempo ne abbiamo abbondantemente, ne userò poco, ma gradirei che non lampeggiasse

i genitori di questi ragazzi non possono essere colpiti dalle sanzioni, ma con l'emendamento intanto introduciamo l'obbligatorietà chiara e scritta per persone che forse arrivano vaccinate, come dice il direttore

Il subemendamento introduce una palese discriminazione tra minori stranieri non accompagnati e quelli accompagnati. Per cui, domando se i diritti e i doveri in ordine alla sanità debbano valere solo per i minori stranieri non accompagnati e non per quelli accompagnati. Al 15 giugno 2017 sono arrivati in Italia 682 minori accompagnati.

si perde il conto) è quello per i minori stranieri; un emendamento del tutto pleonastico perché, come è stato già abbondantemente detto quando il Servizio sanitario nazionale

voto dell'emendamento 1.1500/5, perché lo consideriamo sbagliato nel merito. Ci saremmo aspettati, piuttosto che un bieco accordo sulla base dei minori stranieri, magari una seria presa di posizione da parte della Ministra della sanità sulla salute degli stranieri. *(Applausi dal

Il vigente quadro normativo prevede infatti la loro iscrizione al Servizio sanitario nazionale anche in via temporanea, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 47 del 2017. Di fatto, sono quindi equivalenti a tutti gli altri sottolinearlo in modo più chiaro, secondo me, aiuta meglio la definizione del provvedimento, quindi non si vede motivo per cui l'emendamento non debba essere approvato.

mira semplicemente a eliminare l'obbligatorietà delle vaccinazioni poste nel disegno di legge per un semplice motivo: il decreto-legge in esame è nato

c'è stata l'eradicazione del morbillo in California? Se volete sapere la risposta, è "no". Quindi non è vero che aumentare di un 5 per cento la vaccinazione (e quindi impostarla così) provoca l'eradicazione del morbillo.

considerando che abbiamo sempre puntato sulla raccomandazione, qui noi diciamo: volete farli obbligatori? Gratuiti? Ma li dovete rendere disponibili in modalità monodose, per un'incongruenza del decreto-legge stesso. Il decreto-legge sostiene che, qualora abbiano contratto una patologia per la quale abbiano già sviluppato gli anticorpi e siano immuni, i bambini non sono obbligati a ripetere quel vaccino. Voi non fornite le monodosi, ma, visto che avete fatto una distinzione per l'obbligatorietà esclusivamente caratterizzata da quella che è la produzione delle case farmaceutiche, ossia sono obbligatori l'esavalente (perché viene prodotto l'esavalente), ed è obbligatorio il tetravalente (perché viene prodotto il tetravalente), mi dovete spiegare... Scusate, se una persona ha già avuto il morbillo e non c'è la possibilità di fare la monodose per gli altri tre patogeni, come cavolo si fa a pretendere che le persone si facciano i vaccini? È un'assurdità! *(Applausi della senatrice Serra)*. Se una persona ha già avuto una patologia, il decreto-legge dice che non potete obbligarla a rifare i vaccini. Se non fornite la monodose, come pretendete di vaccinare coloro che hanno già avuto una patologia compresa nell'esavalente o nella tetravalente? Non mi parlate di *ex* articolo 81, perché, se trovate i soldi per far vaccinare in farmacia, dovete dare i vaccini perché questi bambini possano essere vaccinati. Siete degli incompetenti, irresponsabili, incapaci e ingestibili!

presa una decisione: la Presidenza avverte l'Assemblea e gli onorevoli colleghi che il sostegno alla richiesta di voto elettronico sugli emendamenti riferiti a un determinato articolo si intenderà esteso anche agli emendamenti improcedibili, ove ne venga richiesta la votazione. È un modo per semplificare, nel caso di emendamenti improcedibili, salvo che il proponente non ritenga di ritirare l'emendamento. Questa è una decisione assunta precedentemente, quindi non è

È evidente che la richiesta del voto elettronico su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo fa riferimento anche a quelli improcedibili *ex* articolo 81. Essendo coincidente il numero di 15 per i richiedenti il voto elettronico

Signor Presidente, noi facciamo un appello alla Ministra perché questo è un emendamento che aiuterebbe moltissimo, se approvato, anche a svelenire il clima e a fare un'operazione di convincimento, perché molti dei genitori e delle persone che in questo momento sono contrari, spesso lo sono perché vorrebbero avere una sicurezza maggiore e soprattutto un accesso ai Quindi questo emendamento, se approvato, darebbe una mano veramente notevole anche a riaprire un dialogo. Vedo però che la Ministra è presa da altro. Capisco che non abbia interesse: si fanno guerre ideologiche, mentre proposte che invece potrebbero creare un clima diverso, di ragionevolezza

Non si può venire qui a fare interventi di guerra e e poi, quando c'è l'opportunità di poter discutere un emendamento nel merito per poter aiutare la ripresa di un dialogo con le persone e con i genitori che hanno manifestato perplessità, non si vuol sentire.

Presidente, questo emendamento ha una sua validità sotto il profilo scientifico e fattuale, e spiego molto rapidamente il perché. Il decreto-legge prevedeva, originariamente, l'introduzione della obbligatorietà per dodici vaccinazioni. Tra queste 12 vaccinazioni, ce ne sono tre morbillo, parotite e rosolia - che sono state previste esclusivamente per una valutazione, perché esiste il cosiddetto vaccino trivalente. L'emergenza che sta facendo fare una pessima figura all'Italia nel mondo si riferisce al morbillo

il vaccino monocomponente. deve rappresentare non una responsabilità del Governo, ma un impegno dell'Esecutivo a fare in modo che l'industria realizzi, nell'ambito delle proprie discrezionalità aziendali, il vaccino monocomponente. In via alternativa, il Governo può verificare la possibilità che lo faccia lo stabilimento chimico‑farmaceutico di Firenze. Sancire questo principio in termini generali, anche attraverso un ordine del giorno, credo che consenta al Governo di accreditarsi anche di quella maggiore attenzione attenzione e disponibilità che, in qualche occasione, l'Assemblea, a mio avviso non raramente e inopinatamente, sta negando. È questo il motivo per cui invito il Governo a valutare la possibilità di accogliere questa richiesta

ci preoccupa molto, perché siamo convinti che la disponibilità di vaccini monocomponenti sia uno dei tanti strumenti che possono essere messi a disposizione della popolazione per dare l'idea non del pugno duro e della forzatura che lo Stato fa nei loro confronti, ma della flessibilità che garantiamo loro nell'adottare i programmi vaccinali.

Detto questo, credo che forse di questo emendamento si potrebbe richiedere l'accantonamento, così com'è stato fatto per altri, in modo che si abbia una maggiore contezza del perché è stato opposto l'articolo 81.

per tutelare un bene comune collettivo, che è l'equilibrio delle nostre finanze, chiunque governi, siamo chiamati

C'è una prassi, che è bene che tutti i senatori conoscano, in Commissione bilancio, che affida ai Gruppi la possibilità di chiedere un approfondimento da parte del Governo e, quindi, di avere una relazione tecnica

È evidente invece che c'è l'applicazione di un principio di precauzione. Inviterei quindi a raccordarsi i Gruppi delle Commissioni di merito con i Gruppi della Commissione bilancio per eventualmente segnalare alla Commissione bilancio quali sono gli

del senatore D'Ambrosio Lettieri, perché si tratta di monocomponente. La senatrice De Petris ci ha richiamati - e bene ha fatto ad avere in qualche conto quello che sta succedendo fuori: ci sono mamme con bambini Molte di queste potranno anche essere considerate psicolabili, come tutte le mamme eccessivamente preoccupate, ma sono delle cittadine italiane. italiane. Se questo Stato etico, che vuol prendere le mamme per le orecchie e costringerle a vaccinare i propri bambini, potesse avere anche il garbo di venire loro incontro, sedando qualche ansia e preoccupazione, come nel caso dei monodose, non sarebbe male. Ma, signor Presidente, io non vado a guardare nel firmamento, approfitto che c'è il Ministro qua e guardo tra i rovi: i monodose costano di più

voteremo a favore dell'emendamento in esame, anche se preferirei che la senatrice Taverna lo trasformasse in ordine del giorno, perché conosciamo le difficoltà

ovviamente condividiamo questo subemendamento importante, che introdurrebbe i vaccini monodose o monocomponente. Chiedo l'attenzione della relatrice, ma soprattutto del ministro Lorenzin: il comma 2 dell'articolo 1

la possibilità di farli produrre all'Istituto farmaceutico militare di Firenze, non dovendo dare soldi ad aziende estere, producendolo attraverso una struttura statale e guadagnandoci,

Presidente, mi rivolgerei direttamente alla relatrice, se fosse possibile. PRESIDENTE.

rafforzare l'importanza della presenza di formulazioni monocomponente dei vaccini. Avevamo anche valutato che

monocomponente, perché ci rendiamo conto che, in alcuni casi, per recuperare le vaccinazioni, è utile che vi siano; il fatto che non siano così disponibili sul mercato non ci basta, deve essere rafforzata la politica industriale in tal senso. Nel recepire, quindi, tutte le sollecitazioni, chiedo l'accantonamento dell'emendamento

Grazie

che potrebbe rassicurare molti genitori. Stiamo andando verso l'istituzione delle Case della salute. Anzi, qualche Casa della salute è già attiva, per fortuna. Ci sono molti ambulatori

Non capisco che cosa ci sia di tanto strano in tutto questo. Serve semplicemente a dare più tranquillità alle persone che sono lievemente dubbiose.

informate, per aiutarli a dirimere tutti i dubbi, tranquillizzarli ed eventualmente valutare se è il caso di procedere alla vaccinazione del bambino.

Non sappiamo quindi se la senatrice Rizzotti abbia riformulato l'emendamento prevedendo questa condizione solo per i primi sei vaccini e non per i secondi quattro.

Presidente, insisto anche nell'interesse della senatrice Rizzotti, che ha presentato un emendamento

Signor Presidente, vorrei fare una proposta perché ho ben inteso il dubbio espresso dal senatore Arrigoni. Non essendo ancora completata la votazione

La componente Direzione Italia di GAL conferma la propria contrarietà rispetto all'afflittività del sistema sanzionatorio. Invero, durante l'*iter* vi sono state delle modifiche; in particolare, è stata soppressa l'ipotesi sproporzionata della perdita della potestà genitoriale per gli inadempienti. Questo è senz'altro un passo in avanti. Resta ancora da fare qualcosa in più in merito all'afflittività del sistema sanzionatorio sotto il profilo economico, motivo per il quale abbiamo presentato numerosi emendamenti, che hanno ricevuto un parere contrario. Chiediamo inoltre la nostra firma all'emendamento 1.111, se ce lo consente il Gruppo della Lega, per confermare la nostra visione, la nostra posizione e il nostro auspicio.

Presidente, in Commissione siamo stati tutti contrari alle sanzioni. Però è vero che esiste un problema: se noi mettiamo un obbligo e non mettiamo la sanzione, non c'è più l'obbligo.

meccanismo sanzionatorio è qui per primo, perché è il più basso, anch'io mi adeguo a questa sanzione, che è la minima accettabile, e chiedo di

e al Governo, che su questo emendamento ieri hanno espresso un parere contrario: li invito a rivedere il loro parere e a rimettersi all'Aula, visto che, da quanto

Presidente, sono consapevole del fatto che una sanzione è sempre una sanzione, quindi ha un suo effetto negativo. Però bisogna anche essere consapevoli del fatto che, se un dovere, quindi un obbligo, non viene rispettato, il problema di una sanzione si pone. E quando la sanzione è minima, in misura tale da non rappresentare

sanzione pertanto deve avere una sua efficacia, una sua deterrenza e una sua coerenza anche rispetto ai costi generali dell'amministrazione. Altrimenti, guardate, sembriamo una gabbia di pazzi. È vero che molti Parlamenti sfiorano questa situazione, ma cerchiamo di salvaguardare almeno quello italiano. inviterei anch'io i relatori e il Governo a un approfondimento sul tema, quindi o a cambiare giudizio o ad accantonare l'argomento. Senatore Buemi, sono sempre molto attento alle sue argomentazioni, anche perché di solito hanno uno spirito liberale, ma credo che in questo caso lei non abbia colto il problema. Il vero problema problema è che una sanzione molto alta può portare coloro i quali non vogliono i vaccini a pagare e dunque a risolvere il problema. Questo lo può fare una parte della popolazione, se la sanzione è alta, mentre un'altra parte non lo può fare; il che, tra le altre cose, colpisce in maniera selettiva

Visto che quell'altro modo è odioso, forse dovremmo affidarci alla pedagogia e al convincimento, piuttosto che introdurre un elemento di questo tipo. Questa è la ragione per la quale forse varrebbe la pena approfondire questo discorso e arrivare a trovare una soluzione che possa coinvolgere tutta l'Assemblea, perché sarebbe un grande passo in avanti. *(Applausi dai Presidente, io reputo che il senatore Buemi abbia fatto un intervento superficiale e che non consideri

Senatore Buemi, per lei 200 euro non saranno nulla, ma per una famiglia rappresentano la differenza tra riuscire ad arrivare alla fine del mese Stiamo parlando di questo ed è una questione di approccio. È ovvio che c'è una sanzione, ma una sanzione che non tenga conto delle condizioni odierne dei nostri cittadini, significa veramente mettere un capestro odioso al collo delle famiglie, soprattutto nel momento in cui debbono provvedere

Qui, come ha dichiarato la senatrice Petraglia, c'è una vera discriminazione tra chi può e chi non può. Vorrei ricordare al senatore Buemi

Tutti hanno chiesto la rimodulazione, quindi si presume che tutti siano d'accordo con l'idea che le sanzioni, così come previste dal decreto-legge, erano eccessive. Cominciamo a dire questo, perché non c'è un Gruppo che vuole abbassare le sanzioni e altri Gruppi che non vogliono. Così dicendo si fa propaganda e non si dice la verità su com'è andato il dibattito.

Si è cercato quindi un punto di mediazione, che è previsto dall'emendamento 1.112, sul quale ho espresso parere favorevole, che porta le sanzioni pecuniarie da euro 100 a euro 500

In tal senso, voglio anche ricordare - o se preferisce lo faccio successivamente - che, sempre per quanto osservato precedentemente, sull'emendamento 1.112, sul quale mantengo il parere favorevole, va nuovamente riproposta la correzione «di cui al presente articolo» proprio per evitare che si riducano le sanzioni solo ai vaccini previsti dal comma 1 e non a quelli previsti dal comma 1*-ter* nel momento in cui fosse approvato

ma questo decreto-legge si scontra con un macigno che è la conflittualità tra due diritti garantiti dalla Costituzione: il diritto alla salute - ammesso che questa modalità di inoculare vaccini lo sia - e il diritto all'istruzione. Quindi, se introduciamo una sanzione alta, inibiamo il diritto all'istruzione

Coordina la Presidenza, quando può. Quando può, si coordina prima, vista l'esperienza precedente.

tenuta presente nella discussione che stiamo facendo sui diversi articoli ed emendamenti. È ovvio che, se vi è un obbligo vaccinale, ci deve essere anche una sanzione. Siamo consapevoli che tutti i genitori devono essere avvicinati, convinti, aiutati a capire l'importanza della vaccinazione per i propri figli e per tutti i bambini, anche per quelli che non possono assolutamente essere vaccinati e che sono, quindi, in pericolo.

accetta la sanzione da 100 a 500 euro, ma dà la possibilità, a coloro che possono pagare meno, ma anche a coloro che accettano un'educazione sul regime vaccinale,

si rende disponibile a partecipare ad iniziative di informazione previste dall'articolo 2, riceve uno sconto che va dal 50 al 70 al 70 per cento. Abbiamo già comminato la sanzione, abbiamo approvato un emendamento che dice che una persona deve essere aiutata, seguita

potestà genitoriale (poi truffaldinamente diventata responsabilità genitoriale, per una violazione di delega da parte di alcuni Governi fa), non avrebbe mai dovuto esserci. È una delle misure che ha scatenato le reazioni più violente; molti

esprimo un convinto voto favorevole. Esso segna, oltretutto, la convergenza unanime rispetto a un passo in avanti che era stato richiesto sul sistema afflittivo delle

anche il nostro Gruppo ha presentato un emendamento soppressivo del comma 5. La nostra motivazione, però, per la quale voteremo a favore dell'emendamento della Commissione, è parzialmente diversa. Noi chiediamo, infatti, che l'obbligo vaccinale sia giusto e motivato, ma pensiamo che l'introduzione di questi nuovi obblighi e di questo nuovo sistema debba avvenire un po' più gradualmente, con sanzioni meno pesanti all'inizio, sperando che la percentuale dei soggetti vaccinati in Italia in questo modo venga ad aumentare. Se tutto questo non dovesse funzionare, chiaramente si dovrebbe poi tornare a rivedere tutto l'impianto sanzionatorio. Per questo motivo, però, siamo favorevoli alla soppressione del alla revoca della potestà genitoriale, perché riteniamo che questa sia una sanzione, almeno all'inizio, troppo pesante.

anche il Gruppo della Lega Nord voterà a favore della soppressione del comma 5 e quindi a favore di questo emendamento della Commissione che, peraltro, ricalca un nostro emendamento, l'1.143, presentato da noi in Commissione.

Quindi, non c'è contezza di molte malattie infettive, non soltanto quelle comprese nell'obbligo vaccinale, ma parlo di tubercolosi,

che ci allineerebbe ai Paesi più evoluti per quanto riguarda la supervisione delle pratiche vaccinali. In un Paese come il nostro, dove i conflitti di interesse e la corruzione esistono, sarebbe opportuno avere questa struttura. Chiederei di votarlo e cambiare idea sulla sulla volontà di avere qualcuno *super* *partes* che controlla le politiche vaccinali, che non sia quella associazione che avete proposto nel disegno di legge che, però, non corrisponde alle richieste dell'OMS.

Presidente, mi permetta di dire che su questo tema c'è stata una vera e propria tempesta in un bicchiere d'acqua, nel senso che l'impatto del provvedimento sul sistema sarà particolarmente rilevante, come è facile immaginare. possibilità, anche in relazione a quanto espressamente previsto dall'articolo 11 della legge n. 69 del 2009 e dei conseguenti decreti attuativi che hanno disciplinato la farmacia dei servizi, avrebbe potuto

vaccinali che sarebbero stati affiancati, dalle attività svolte negli ambulatori dai medici di medicina generale e in parte anche dalle farmacie. Ho sentito delle polemiche fuori luogo. Mi consenta di esprimere il mio garbato deploro rispetto a questo atteggiamento di considerare come inopinatamente ben sei formulazioni di emendamenti, scritti anche da penne particolarmente competenti, hanno subito la ghigliottina della Commissione bilancio. A tale proposito vorrei esprimere per il garbo e la cortese disponibilità che il presidente Tonini ha offerto all'Assemblea in relazione all'attività posta in essere dalla Commissione che brillantemente presiede. Sulla base di queste considerazioni certamente accolgo con favore il pensiero della relatrice di recuperare un parere positivo sull'ordine del giorno G1.300, ma esprimo la mia profonda delusione

tra Forza Italia e Partito Democratico cui abbiamo assistito da ieri sulla possibilità di effettuare le vaccinazioni presso le farmacie pubbliche e private del territorio del territorio con i medici e gli infermieri. Ci sarebbe tanto da discutere, ma il tempo è pochissimo. Sarebbe infatti interessante capire se i medici e gli infermieri sono quelli del Servizio sanitario nazionale, se verranno assunti

un presidio sanitario previsto dal nostro regolamento e dai nostri ordinamenti, ha una lunga storia e già presta presta servizi importanti di primo soccorso e tutti i servizi inerenti alla persona, tra cui anche alcune piccole prestazioni di tipo sanitario. E lo fa assolutamente in sicurezza, con farmacisti che sono assolutamente laureati e, nella fattispecie della questione vaccinale, con professionisti, quindi con infermieri e medici, che sono titolati a fare questo. Vorrei anche ricordare che, proprio perché le farmacie sono capillari su tutto il nostro territorio nazionale, come nel caso delle famose farmacie rurali, queste prestano un servizio importantissimo *in loco*; quindi aiuterebbero anche le famiglie a non doversi spostare nel centro urbano, dove certamente,

collabora fortemente con le aziende sanitarie delle ASL e con il Servizio sanitario nazionale. Pertanto ci auguriamo

mi associo alle valutazioni che ha fatto la collega Petraglia e quindi non insisto. Vorrei però sottolineare un ulteriore elemento che considero deplorevole (per usare un termine appena utilizzato). Mi riferisco al fatto che non sia stata richiesta la formula di rito: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare». Lo dico in termini economici, perché chiaramente questo è un tipo di impegno che

il Governo non dovrebbe - a mio avviso, ma non mi permetto di rivolgere un suggerimento diretto - adottare un impegno di questo tipo, senza la formula di rito, che è motivata dal rispetto dell'equilibrio di bilancio che qui viene violato, pur essendo un principio costituzionale.

ordine del giorno. Ricordo a tutti i colleghi che già prima di questo decreto-legge c'era l'obbligo di vaccinazione, sia pure per un numero di vaccini inferiore. Pertanto, rendere più agevole la vita agli italiani che magari vivono in zone

a favore, ma faccio presente che in Commissione sanità era stato formulato un emendamento più preciso più preciso in cui il Ministro si impegnava, con un decreto ministeriale, a dettagliare le modalità. Faccio presente che è importante la presenza del medico, che non è convertibile l'infermiere con il medico ed è importante redigere il certificato di vaccinazione e inviarlo alle ASL, in modo che vengano aggiunte la vaccinazione e gli eventuali effetti collaterali all'Anagrafe nazionale che si è predisposta.

Signor Presidente, sono molto d'accordo sulla farmacia dei servizi. Ho sempre visto il farmacista come un alleato e non come un nemico,

Se è vero che questo servizio può essere svolto nelle farmacie, non vedo perché non possa essere fatto in presenza di medici e di infermieri

Signor Presidente, ho ascoltato alcuni interventi che facevano riferimento ad accordi. Siccome erano riferiti anche al contesto nel quale si svolgeva la discussione su un emendamento che avevo sottoscritto, vorrei sottolineare, con grande fermezza e chiarezza, che il rapporto che la componente Direzione Italia mantiene con il PD è dialetticamente corretto, trasparente, ma, naturalmente, di ferma e netta opposizione rispetto a posizioni divergenti su tanti aspetti. Voglio evidenziarlo perché

Signor Presidente, esprimo la mia più convinta e determinata vicinanza e solidarietà a Paolo Berizzi, cronista di «la Repubblica», vigliaccamente minacciato dai fascisti. Sappia Berizzi che non è solo nella sua coraggiosa ricerca della verità e nella sua attività di informazione sui rigurgiti passatisti e violenti che infestano il Nord d'Italia. Abbiamo sindaci di centrodestra che nominano neonazisti assessori, concessionari di beni pubblici che trasformano spiagge in sedi di associazioni per delinquere e deputati sanbabilini che insultano colleghi in modo irripetibile. Berizzi continui a raccontarci queste cose e a renderci vigili; ha tutto il nostro sostegno. E sappia questa gentaglia che alimentarsi di ignoranza e di arroganza non li farà prevalere, perché i valori della democrazia e della libertà sono più forti.

Vede, Presidente, nel mio Paese, a Tradate, negli scorsi giorni è accaduto un fatto abbastanza grave. Due richiedenti asilo che hanno già ottenuto il diniego del permesso di essere riconosciuti come profughi si sono azzuffati ponendo in essere atti di vera violenza. signor Presidente, il prefetto di Varese ha emesso un provvedimento che mi lascia abbastanza basito. Scrive il perfetto nel suo provvedimento: atteso che tale condotta è pregiudizievole nei confronti del percorso di integrazione e prova del rifiuto da parte dei suddetti - ci sono nomi e cognomi e anche cittadinanza e provenienza, quindi tutti ovviamente identificati - identificati - di accettazione delle normali, minime, imprescindibili regole che devono essere rispettate per la convivenza in ambito collettivo, integra gli estremi di una condotta gravemente violenta che ha determinato un danneggiamento dei beni del CAS. Presidente? Ci si aspetterebbe l'espulsione dal Paese. No. La fine di questo percorso è semplicemente: ordina l'immediato allontanamento dal centro di accoglienza. È chiaro che si crea un paradosso perché chi rispetta le regole